Grazie

c'è piena apertura e trasparenza da parte della Difesa, documentando e rendendo disponibile in rete tutta la documentazione tecnica in possesso. Sul sito ufficiale della Marina militare, alla voce "bandi di gara", è possibile accedere ai dati relativi alle analisi dell'acqua dell'*ex* reattore prima del trattamento, mentre le risultanze degli esami dopo il trattamento sono state fornite dal CISAM alle istituzioni locali di Pisa e di Livorno (Comune, Provincia, prefettura), oltre che all'ISPRA e all'ASL, nonché all'Agenzia regionale per la protezione ambientale Toscana che le ha pubblicate integralmente sul proprio sito. Venendo al tema posto dall'interrogante, il reattore di ricerca a piscina Galileo Galilei, presso il Centro interforze studi e applicazioni militari (CISAM) di San Piero a Grado, ha definitivamente cessato l'attività nel 1980 negli anni seguenti sono state condotte in assoluta sicurezza, secondo le procedure più idonee, tutte le operazioni di *decommissioning* dell'impianto. Nel 2010 è stato completato lo smantellamento del circuito di refrigerazione secondario e delle barre di controllo ed è iniziata la procedura di smantellamento della piscina, suddivisa in quattro fasi. La fase uno (eliminazione dell'acqua della piscina e condizionamento del materiale presente) si è conclusa nel maggio 2015 con il rilascio delle certificazioni, da parte dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dello stato ambientale del sito. La fase due, attualmente in corso, prevede lo smantellamento del circuito primario, dell'impianto di purificazione attiva, dell'impianto raccolta effluenti liquidi radioattivi e dei drenaggi e comporterà la realizzazione di circa centotrenta contenitori di rifiuti radioattivi a bassa e media attività, ovvero che perdono quasi completamente la loro radioattività nell'arco di quasi un secolo. e quattro - ancora oggetto di studio - comprendono, al momento, interventi sugli impianti ausiliari e sulla struttura in cemento armato della piscina e consentiranno il completamento della procedura di smantellamento della piscina. Con riferimento, invece, alla quantità di rifiuti radioattivi che sarà prodotta durante tali ultime due fasi, non è possibile fare una stima attendibile, in quanto il dato dipenderà in larga misura dall'effettivo stato radiologico dei componenti che potrà essere verificato solo in corso d'opera. Ad oggi, nel deposito del CISAM sono temporaneamente conservati 1.140 contenitori di rifiuti radioattivi condizionati derivanti da attività della Difesa. Per quanto riguarda i rifiuti radioattivi prodotti dagli ospedali militari, si precisa che, in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto radioattivo da trattare (quantità, tipologia di isotopi e attività), vengono messe in atto le misure di radioprotezione determinate dall'esperto qualificato dell'ente (responsabile della protezione dei lavoratori dal rischio radiologico), che prevedono anche le modalità di smaltimento degli stessi. Ogni struttura sanitaria gestisce tali rifiuti con ditte specializzate di settore - sulla base di apposite convenzioni - che provvedono alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti in accordo alla vigente normativa. Per quanto concerne la possibilità di smaltire nel Deposito nazionale di rifiuti radioattivi, come precisato dall'interrogante, a «titolo definitivo anche i rifiuti radioattivi prodotti da attività afferenti al Ministero della difesa», si segnala che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, interessato al riguardo, ha comunicato che, in linea con gli articoli 11 e 12 della direttiva 2011/70/Euratom, il Programma nazionale di gestione del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi predisposto dai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico - in fase di valutazione ambientale strategica (VAS) - prevede, allo stato, soltanto la gestione dei rifiuti derivanti da attività civili. Quanto, infine, alle attività di sorveglianza e di controllo delle operazioni di smantellamento, la Difesa si è avvalsa, nella prima fase dello smantellamento, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), deputato a tali attività in ambito civile, mentre le analisi delle acque trattate e delle matrici ambientali sono state eseguite, oltre che dal CISAM, dall'ENEA, assicurando così una condizione di terzietà e garanzia. Anche nel corso della seconda fase saranno effettuati controlli a campione da parte dell'ISPRA e dell'Università di Pisa.

in cui vengono smaltiti i rifiuti in questione. Abbiamo appena sentito che il Programma nazionale, che tra l'altro è ancora in corso di definizione, prevede lo smaltimento nel Deposito unico nazionale

questo Governo è fortemente in ritardo proprio in merito al primo passo, il fondamento di tutta la gestione del processo di smaltimento, di *decommisioning* che è la redazione del Programma nazionale.

Quindi, non sappiamo effettivamente che cosa verrà fatto in seguito per completare la procedura di smaltimento.

addetto a sovraintendere alle procedure di *decommissioning*, anche se siamo i primi a dire che è stato nominato un direttore che non è in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi. Per tutti questi motivi, non posso ritenermi soddisfatto.

in premessa ritengo necessario sottolineare che concordiamo sull'importanza della bachicoltura italiana, tanto che abbiamo un'unità specializzata per la ricerca in questo campo del nostro ente di ricerca (CREA). Nel merito delle questioni sollevate dall'interrogante devo purtroppo ricordare che, nell'ambito del nuovo corso della politica di aiuto comunitario, adottata dall'Unione europea nel giugno 2013, l'aiuto a favore dei bachicoltori precedentemente riconosciuto non è stato confermato. Sul fronte dell'aiuto accoppiato, poi, l'attuale suddivisione è stata frutto di un elaborato percorso di condivisione con le Regioni, le Province autonome e le organizzazioni agricole, per raggiungere un risultato concreto di sostegno ad alcune produzioni nazionali. Per la revisione di medio termine dell'aiuto accoppiato, prevista dalla regolamentazione europea, si è condiviso con gli stessi soggetti di apportare semplici aggiustamenti nei *plafond*, fermi restando i settori da sostenere. In tal senso, lo scorso 1° agosto abbiamo notificato quanto concordato alle competenti autorità europee. Resta però l'importanza del tema proposto e che potremo sollevare in sede europea - e in questo concordiamo pienamente con l'interrogante - anche in vista della costruzione della prossima riforma della politica agricola comune. [DALLA

riprendendo quota, perché anche l'impresa serica chiede con forza la qualità del prodotto; qualità che in altri Paesi produttori, per prima la Cina, non viene espressa per la nostra industria. Quindi, accolgo positivamente

soddisfatto della risposta e soprattutto dell'impegno del Vice Ministro.

al Senato della Repubblica, di fronte alla Presidenza, mentire. L'interpellanza di oggi, che riprende quella del 13 ottobre, parla della Autorità nazionale competente per l'attività regolatrice dei farmaci in Italia, ente di diritto pubblico che opera in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia, secondo l'indirizzo del Ministero della salute e sotto la vigilanza dei Ministeri della la determinazione del prezzo dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale avviene mediante la contrattazione tra l'Aifa e le aziende farmaceutiche

Quindi, la procedura negoziale sulla fissazione del prezzo dovrebbe essere condotta sulla base di criteri ed elementi tra i quali sono da tenere in massima considerazione la trasparenza, l'utilità del nuovo medicinale per la prevenzione o il trattamento di patologie o di sintomi rilevanti nei confronti dei quali il medicinale ha una sua efficacia. Si devono tenere presenti i volumi di vendita, che dovrebbero essere ipotizzati in base ad una stima la più accurata possibile, possibile, fondata sui dati scientifici ed epidemiologici aggiornati e disponibili al momento della negoziazione. Questa è la parte del discorso di carattere generale: adesso c'è il dramma.

L'AIFA, con il suo presidente Pani, avrebbe assunto una "trattativa secretata" con l'industria farmaceutica: in sostanza, un'agenzia di diritto pubblico tratta con una società americana, la Gilead, in maniera segreta sul prezzo che, invece di garantire un prezzo accessibile al farmaco, si sarebbe conclusa con la determinazione di un altissimo costo del farmaco, tale che un ciclo di cura completo costa poco meno poco meno di 40.000 euro per paziente, con un effetto molto negativo sulla spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale, che vira sempre di più verso

al contrario di quanto avviene in Egitto e in India, divenute mete per gli italiani di "turismo terapeutico" che - a giudizio dell'interrogante - è ancor più atroce del turismo sessuale, che In Egitto, ove il farmaco è in concessione dalla stessa Gilead - è lo stesso prodotto, conservato nella stessa scatola - con l'accordo stipulato tra il Ministro

È causa di cirrosi epatica per il 35 per cento degli affetti; porta a emorragie del tratto gastroenterico per varici esofagee; porta ad ascite e a cirrosi e porta dall'1 al 4 per

Tutti gli osservatori epidemiologici nazionali più qualificati (Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità; istituto nazionale di malattie infettive Spallanzani di Roma; progetto Dionysos), all'epoca della contrattazione del prezzo di Sovaldi,

costo del farmaco sulla salute pubblica e sulla stessa sopravvivenza di centinaia di migliaia di pazienti sarebbe urgente istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla negoziazione del prezzo del Sovaldi, affinché si faccia definitivamente chiarezza chiarezza sull'incredibile vicenda della trattativa riservata e secretata per verificarne l'equità e la correttezza. Io stesso mi sono rivolto al Ministero dell'economia e delle finanze per chiedere il suo intervento.

di rinforzo della prima. Giustamente lei ha detto che anche nel 2006 e 2007 gli è stato dato, ma i 2.000 euro nel 2006 e 2007 non sono i 70.000 euro di adesso.

le tessere di Comunione e Liberazione. Ma - mi scusi - è un movimento che si autodefinisce ecclesiale e non fa tessere. Quindi, non può venire qui a dirci che sono estranei perché non hanno

avrebbe perduto nella causa di ricorso al TAR promossa da altro concorrente, AIFA l'ha trasferito con una manovra incredibile ad altro incarico, in modo da delegittimare il ricorso stesso: un gioco a tre carte

espletare le normali attitudini della vita. Noi gli stiamo vicini, vicinissimi. Come eletto in Consiglio regionale è il popolo che decide, ma in un'agenzia con le pressioni menzionate il presidente che va a fare il direttore generale non assicurare trasparenza, soprattutto quando la Conferenza Stato-Regioni è convocata per la prossima settimana.

di vista, le cose vadano viste con una certa serenità, legalità e trasparenza.

abbia fatto lievitare notevolmente il prezzo contrattato dai vertici AIFA con la Gilead nella negoziazione del farmaco e se tale sottostima, in dispregio a tutti i dati epidemiologici all'epoca disponibili, non possa configurare anche ipotetici profili di dolo.

e quindi fruibili in qualsiasi momento, forniti dalla stessa Agenzia italiana del farmaco. In via preliminare occorre evidenziare che le questioni sollevate dal senatore Barani coinvolgono ambiti diversi della regolamentazione del mercato farmaceutico. A tale riguardo, si sottolinea che il settore in questione è caratterizzato da un elevato livello di regolamentazione da parte di fonti normative sia europee che nazionali. In tal senso, le attività dell'AIFA, per quanto attiene all'ambito regolatorio, sono sicuramente - mi permetterei di segnalarlo - coerenti con l'assetto normativo comunitario e nazionale. In particolare, la determinazione del prezzo dei farmaci

la negoziazione del prezzo di una nuova specialità medicinale avviene secondo i seguenti criteri: rapporto costo/efficacia positivo: il medicinale è ritenuto utile per il trattamento di patologie per le quali non esiste alcuna terapia efficace, o fornisce una risposta più adeguata rispetto a farmaci già disponibili per le medesime indicazioni terapeutiche; rapporto rischio/beneficio più favorevole rispetto a farmaci già disponibili per le stesse indicazioni; valutazione dell'impatto economico sul Servizio sanitario nazionale; miglior rapporto costo terapia per giorno a confronto con prodotti della stessa efficacia; stima delle quote di mercato acquisibili; confronto con i prezzi e i consumi degli altri Paesi europei. Questi erano i criteri della delibera CIPE. Nella valutazione dell'efficacia e del prezzo di un farmaco, l'AIFA si avvale del supporto della commissione tecnico-scientifica

L'*iter* relativo alla procedura di prezzo e di rimborso definito in termini generali dalla citata delibera CIPE si articola in una serie di fasi che sono disciplinate, nella loro tempistica, anche dal regolamento AIFA per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'accesso ai documenti amministrativi e per la dematerializzazione 1° settembre 2010, e dallo stesso regolamento della commissione tecnico-scientifica e del comitato prezzi e rimborsi. Gli strumenti utilizzati dall'Agenzia, quale autorità nazionale competente per la fissazione dei prezzi, permettono di ottenere le condizioni economiche e di accesso ai farmaci tra le più favorevoli, in relazione alle caratteristiche dello specifico contesto territoriale considerato, che è dato riscontrare tra i Paesi europei. Ciò comporta, talune volte, l'esigenza di mantenere la riservatezza sull'effettivo prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale per i medicinali oggetto di negoziazione, non ponendosi tale modalità

è, nelle ipotesi specifiche in cui tali accordi possono intervenire, un utile strumento per assicurare la possibilità di far valere le peculiarità del singolo prodotto nel contesto nazionale nel confronto con l'azienda che si accinge a immettere il proprio farmaco sul mercato e ottenere addirittura condizioni economiche più favorevoli per il nostro Servizio sanitario nazionale. Svolte queste considerazioni - che mi sembravano utili e in coerenza con tutte le osservazioni che ha fatto il senatore Barani - con riferimento al caso in esame AlFA ha negoziato un accordo contrattuale per la definizione del prezzo per il farmaco per la cura dell'epatite C e la conseguente presa in carico dei pazienti affetti da HCV, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, e tale accordo è attualmente oggetto di nuova contrattazione per sopravvenuta scadenza temporale del precedente. È ad ogni modo importante sottolineare che ad oggi oltre 50.000 pazienti affetti da epatite C sono stati già trattati, con integrale imputazione dei relativi costi al Servizio sanitario nazionale. È infatti importante rilevare che l'Italia resta uno dei primi Paesi europei ad aver avviato il procedimento di negoziazione del prezzo del Sofosbuvir, con l'obiettivo di individuare le migliori condizioni per la rimborsabilità dello stesso a carico del Servizio sanitario nazionale. Il nostro Paese, dunque, si caratterizza per i prezzi dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale e la spesa farmaceutica *pro capite* capite* più bassi rispetto agli altri Paesi europei; tale affermazione resta valida anche nel caso specifico qui trattato di contrattazione del prezzo dei farmaci con la Gilead, che infatti risulta il più contenuto - conferma AIFA - nel contesto europeo. Il nostro è un sistema che, garantendo cure di qualità a tutti con costi a carico del sistema sanitario, è costantemente posto di fronte alla sfida di combinare

il massimo beneficio, garantendo al contempo la sostenibilità del sistema e l'equità e l'omogeneità dell'accesso stesso, è stata senza dubbio un'esigenza prioritaria che l'Agenzia ha perseguito e continua a perseguire con determinazione ed impegno massimi, condividendo le priorità anche con le associazioni dei pazienti cui la cura è destinata. Va inoltre ricordato che, con l'articolo 1, comma 593, della legge di stabilità per il 2014, è stato istituito, presso il Ministero della salute, un Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi, con uno stanziamento da parte dello Stato di 100 milioni di euro per il 2015

Il Ministro della salute ha fortemente voluto la costituzione del summenzionato fondo, proprio al fine di consentire il trattamento dei casi che presentano requisiti di maggiore urgenza. Per un approccio efficace al problema, sarà tuttavia necessario avviare una nuova riflessione, più ampia, che preveda un confronto e una collaborazione che noi auspichiamo addirittura a livello comunitario, quindi europeo. che era già emersa, proprio su impulso dell'Italia, durante il semestre europeo di Presidenza italiana. In tale sede e in occasioni successive si è discusso concretamente dell'opportunità di una procedura di negoziazione addirittura su scala europea, che possa far valere il peso dei grandi numeri, pur nel rispetto delle differenze di approccio che ogni singolo Stato può avere sulla materia. Si tratta certo di un progetto ambizioso, che presuppone la condivisione di dati e di esperienze, nonché la disponibilità a convergere su soluzioni comuni per i Paesi membri. Finché dunque non saranno concordate a livello europeo nuove norme che consentano di differenziare i termini della contrattazione sulla base di elementi come la prevalenza di una patologia e le caratteristiche dei singoli mercati farmaceutici, l'azione delle agenzie regolatorie (quindi di AIFA) e, più in generale, dei servizi di sanità pubblica nazionali sarà comunque vincolata da un complesso di norme, spesso di fonte sovranazionale, che delimitano gli ambiti di autonomia nazionale e che proteggono trasversalmente - com'è noto - i diritti di proprietà industriale, con norme sui brevetti che garantiscono in alcune circostanze le aziende titolari nell'intero contesto dell'Unione europea e addirittura anche oltre. Il compito delle autorità nazionali preposte alla tutela della salute pubblica consiste dunque in una continua e difficile opera di bilanciamento tra la primaria esigenza di garantire, da un lato, il miglior trattamento sanitario possibile ai propri cittadini con un oculato impiego delle risorse disponibili e, dall'altro, la tutela dei legittimi diritti delle aziende che hanno investito in sperimentazione e ricerca, cercando di svolgere al contempo un'importante funzione di stimolo nei confronti dell'industria

normativamente coerente con gli obiettivi di salute pubblica e proporzionata alla portata delle prerogative che la legge attribuisce all'Agenzia. Da ultimo, non mi sembra

in materia di trasparenza sugli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche, che in estrema sintesi, impegna il Governo, per il futuro, ad evitare accordi di riservatezza, ad eccezione di casi straordinari motivati dalla rilevanza terapeutica e dalle dimensioni dell'impatto finanziario - valutando comunque, anche in tali specifiche circostanze, di conformarsi agli orientamenti comunitari

Questi farmaci innovativi sono andati in prevalenza al Nord. Non è giusto e non è corretto. Non è così che si uniforma la sanità in Italia. Lei ha parlato di *pay back*. Ma lo avevo già detto io

prima di entrare nel merito degli altri quesiti posti, si forniscono alcune precisazioni con specifico riguardo all'allestimento, da parte di AIFA, di un proprio *stand* nell'ambito del Meeting di Rimini del movimento Comunione e Liberazione. Pur avendo già fornito chiarimenti in proposito, proprio in quest'Aula, lo scorso 13 ottobre, ribadisco ancora una volta, e tutte le volte che sarà ancora necessario, che l'allestimento di uno *stand* di AIFA alla manifestazione fieristica

Invero, AIFA riferisce che la scelta di allestire un proprio spazio espositivo nell'ambito della predetta manifestazione va inquadrata in una precisa politica di investimento in attività di informazione e promozione, finalizzata a dare adeguatamente conto dell'impegno quotidiano portato avanti dall'Agenzia a tutela della salute pubblica. Al fine di procedere all'allestimento dello spazio espositivo, si è proceduto con regolare richiesta di acquisto all'Ufficio affari amministrativi, contabilità e bilancio; richiesta che è stata successivamente integrata da una relazione esplicativa delle ragioni alla base della scelta. La legge istitutiva dell'AIFA e il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale AIFA prevedono che il direttore generale, legale rappresentante dell'Agenzia, sia l'organo cui competono i poteri di gestione e di direzione. Alla nomina del direttore generale si procede con decreto del Ministro della salute, in qualità di organo vigilante e con funzioni di indirizzo dell'Agenzia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

il Ministro della salute un contratto di lavoro avente durata quinquennale a decorrere dalla nomina. Il suddetto contratto disciplina l'incarico ed il relativo trattamento giuridico ed economico. Ciò premesso, al fine di fornire una chiara ed esaustiva risposta ai quesiti dell'interrogante è necessario procedere ad una puntuale ricostruzione delle questioni. Con determina del direttore generale n. 792 del 24 luglio 2014, era stato istituito presso l'AIFA un gruppo di lavoro incaricato di accertare

All'esito della disamina della normativa succedutasi negli anni, il gruppo di lavoro istituito ha evidenziato che, da un punto di vista formale, i compensi che il direttore generale dell'AIFA percepisce per l'incarico di rappresentante italiano presso il CHMP provengono sicuramente dal bilancio dell'Agenzia e non direttamente dall'EMA. Tuttavia, da un punto di vista sostanziale, tali compensi hanno origine comunitaria e vincolo di destinazione immodificabile. Si è così ritenuto decisivo, ai fini dell'accertamento richiesto, verificare se nella nozione di «compensi a carico delle pubbliche finanze» rientri ogni somma che confluisca nel bilancio di una pubblica amministrazione, indipendentemente dalla provenienza della stessa o dall'esistenza di un vincolo di destinazione (com'era per quei Il gruppo di lavoro ha evidenziato come non sia rinvenibile alcuna disposizione normativa e/o documento interpretativo della nozione di «pubbliche finanze» che possa in qualche modo far propendere per una soluzione piuttosto che per un'altra. Alla luce di tali considerazioni, il gruppo di lavoro ha ritenuto di propendere per un'interpretazione della norma che definisce il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, nel senso che la stessa deve ritenersi riferita ai compensi percepiti a carico delle finanze pubbliche e, per tale ragione, non è direttamente applicabile agli emolumenti di diversa provenienza, tra i quali rientrano i compensi derivanti dall'EMA. Nella seduta del 30 gennaio 2015, il consiglio di amministrazione dell'AIFA, esaminate le risultanze del summenzionato gruppo di lavoro, ha ritenuto opportuno investire della questione i Ministeri vigilanti, al fine di ottenere indicazioni che consentissero di superare i riscontrati dubbi interpretativi e di applicabilità. I pareri resi sul punto dai Ministeri vigilanti hanno evidenziato, ad onore della ricostruzione storica, posizioni tra loro contrapposte. Pertanto, all'esito della seduta del consiglio di amministrazione del 29 luglio 2015, il presidente del consiglio di amministrazione ha indirizzato al Ministero della salute apposita nota finalizzata a valutare l'opportunità di richiedere un parere parere in merito all'Avvocatura generale dello Stato. Di tale iniziativa il presidente del consiglio di amministrazione informava con nota del 31 luglio 2015 i componenti del consiglio di Nella seduta dell'8 settembre 2015, il consiglio di amministrazione ha ritenuto di sospendere ogni determinazione sull'argomento, in attesa di conoscere gli esiti degli approfondimenti richiesti al Ministero della salute, e, al contempo, di non procedere ad alcun pagamento dei compensi in questione. In data 3 dicembre 2015, l'Avvocatura generale dello Stato ha reso la consultazione richiesta dal Ministero. Nel parere, l'Avvocatura generale dello Stato ha sottolineato come «il quadro appare complesso e non univocamente definito, il che può naturalmente avere ingenerato equivoci o false consapevolezze anche in capo agli interessati, con l'ovvia conseguenza che eventuali provvedimenti di recupero delle somme eccedenti il tetto retributivo peraltro sinora corrisposte dallo stesso datore di lavoro sarebbero probabilmente forieri probabilmente forieri di contenziosi dall'esito alquanto incerto». In data 18 dicembre 2015, il coordinatore dell'area amministrativa dell'Agenzia, preso atto dei contenuti del parere dell'Avvocatura, ha revocato la sospensione del pagamento degli emolumenti; sospensione, che lo stesso coordinatore dell'area aveva disposto, in autotutela, con precedente nota del 10 novembre 2015. Il 29 aprile 2016, a seguito di specifico rilievo sollevato dal collegio dei revisori, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha approvato il bilancio consuntivo dell'Agenzia, prevedendo la modifica del fondo rischi mediante l'introduzione della voce dei costi «debiti verso l'erario», e ha disposto la contestuale apposizione di una voce in contropartita alla voce «altri ricavi», relativa ai crediti per nota di addebito da emettere nei confronti del direttore dell'AIFA. Durante la seduta del 13 maggio 2016, a seguito della richiesta dei consiglieri circa l'andamento della richiesta del recupero delle somme da trasmettere ai componenti CHMP, il presidente ha informato il consiglio che erano in corso le opportune verifiche interne per individuare il responsabile del procedimento che avrebbe effettuato questo avrebbe effettuato questo recupero. Giova a questo punto evidenziare che il 17 giugno 2016, il vice procuratore generale della Corte dei conti ha comunicato che l'istruttoria, aperta su segnalazione del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, relativa ai compensi attribuiti ai rappresentanti italiani presso il CHMP «è stata archiviata allo stato degli atti», dando atto che «il quadro

pareri resi sull'argomento, così che non si è ritenuto di ravvedere profili gravemente colposi rispetto alle decisioni assunte in ordine all'erogazione dei compensi». Sempre nel mese l'Agenzia ha valutato l'opportunità di emettere apposite note di addebito in relazione alle somme eccedenti il limite di cui all'articolo 23-*ter*, partendo dalla considerazione che il professor Pani, nel suo ruolo di direttore generale dell'Agenzia e al contempo di membro del CHMP,

oculi* la competenza funzionale di avviare e gestire il procedimento di emissione delle note di addebito nei confronti di soggetti che non siano dipendenti dell'Agenzia.

che il compito di emettere la nota non avrebbe potuto essere esercitato da quest'ultimo per l'esistenza di un evidente conflitto di interessi. Si è dunque ritenuto opportuno rimettere la questione al Ministero della salute, al fine di di acquisire chiarimenti circa la necessità e la corretta modalità di avvio del procedimento. Il Ministero ha ritenuto opportuno richiedere un nuovo parere dell'Avvocatura generale dello Stato

si inserisce l'iniziativa del dirigente dell'area coordinamento affari amministrativi, contabilità e bilancio, che in data 29 agosto, inviava al direttore dell'AIFA nota di debito, *ex* articolo 1219 del codice civile. Quanto alla specifica questione relativa alla posizione lavorativa del dottor Torre, osservo quanto segue: in data 11 luglio 2016, in attuazione dell'articolo 32 del Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale AIFA, è stato dato avvio al procedimento per il conferimento di posti di funzione dirigenziale di livello non generale, venendo meno, per effetto della riorganizzazione, gli incarichi assegnati. Agli esiti della selezione dei *curricula*

al nuovo regolamento, le funzioni dell'ufficio contabilità e bilancio sono state ricollocate nel quadro delle nuove disposizioni. In data 1° agosto 2016 la stessa direzione generale di AIFA ha tempestivamente comunicato all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, istituto di provenienza del dottor Torre, affinché si attivasse a far cessare il comando dello stesso. Tenuto conto dei fatti, così come faticosamente, dettagliatamente e cronologicamente ho voluto appare quindi, anche in questo caso, non corretto parlare di «revoca unilaterale» del comando del dottor Torre o di allontanamento dello stesso da parte dell'Agenzia, correlandola alla nota di addebito ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile. Dall'esposizione dei fatti, emerge con evidenza come le azioni poste in essere dal presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, siano state tempestive e volte alla risoluzione del problema nel momento in cui lo stesso si è manifestato. sottolineare come, sia nel parere dell'Avvocatura generale dello Stato che nella notifica informativa di avvenuta archiviazione della Corte dei conti, il quadro giuridico sotteso a questa complessa vicenda di recupero viene definito, per per l'appunto: «complesso e non univocamente definito» ed anche particolarmente difficile nella sua interpretazione.

generale. Il consiglio di amministrazione di AIFA, a seguito di una segnalazione del collegio dei revisori dei conti e di due pareri espressi dalla Ragioneria generale dello Stato, si accorge che questi, invece di 240.000 euro l'anno, percepiva 500.000 euro.

Costui, dopo tutte le delibere, dà esecuzione a quanto deliberato e, per lesa maestà, viene cacciato dall'AIFA, perché, come giustamente si è detto, era un distaccato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

consiglio di amministrazione

perché dicono che percepire 90.000 euro l'anno di stipendio base è troppo, anche se è agganciato al reddito di un primo giudice di Cassazione e c'è un direttore generale che prende 500.000

anche a bilancio nel 2015. Perché cacciare quello che «intempestivamente» ha notificato la nota di debito al dottor Pani, nonostante questa fosse stata trasmessa quattro mesi dopo la delibera votata all'unanimità dal consiglio di amministrazione presieduto da Melazzini?

Chi le ha preparato la risposta ha cercato di confonderla, mentre io l'ho detta in termini più comprensibili, come le dico in termini più comprensibili che l'AIFA è un'agenzia che non deve promuovere niente. non deve promuovere niente. Non deve spendere niente per la promozione di se stessa. Non deve finanziare nessuno. Deve controllare e impedire che le industrie farmaceutiche se ne approfittino e impediscano la cura agli ammalati. Deve fare solamente questo.

Chinè e il Ministro le cose le sapevano e dopo una delibera del consiglio di amministrazione non si può fare il gioco delle tre carte per far sì che non vengano restituite somme indebitamente prese, ancorché in maniera certamente non dolosa, né colposa. È stato un errore e agli errori, come ha detto, la Corte dei conti bisogna porre

mediante gli atti di sindacato ispettivo in discussione, il senatore Lo Giudice sottolinea - nel contesto anteriore al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari - le esigenze dei Comuni in relazione alla liquidazione dei contributi riferibili alle annualità pregresse, dovuti per effetto della legge n. 392 del 1941. Al fine di risolvere le criticità rilevate, nella medesima prospettiva delineata dall'interrogante, la legge di stabilità per il 2015 ha, come noto, radicalmente innovato la disciplina delle funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, offrendo l'opportunità - una volta fronteggiata l'emergenza - di costruire un nuovo modello di maggiore efficienza, equità e risparmio economico. Il Ministero della giustizia ha assunto, sin nell'immediatezza, una serie di iniziative preparatorie, con la finalità di agevolare l'indifferibile trasferimento di funzioni, previsto ed effettivamente entrato in vigore dal 1° settembre 2015, adottando nuove misure organizzative tese a garantire la continuità dei servizi e dell'attività giurisdizionale. Nella prospettiva di raccogliere, attraverso il metodo del confronto, i contributi dei soggetti coinvolti dall'attuazione del nuovo modello di gestione, è stato istituito un tavolo tecnico permanente, aperto alle amministrazioni interessate, per la coerente definizione degli indirizzi politici delle amministrazioni centrali e per il monitoraggio delle attività necessarie alla relativa e coerente attuazione. È stata, in particolare, avviata e consolidata una proficua interlocuzione con gli enti istituzionali coinvolti, in special modo con l'ANCI, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, grazie alla quale si è pervenuti all'adozione congiunta di una convenzione quadro, sperimentando la praticabilità di forme di collaborazione tra amministrazione centrale e amministrazioni periferiche in termini di assistenza nonché di supporto. È stato, inoltre, adottato il Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 2015, che assume la peculiare funzione - nel quadro generale consegnato dalla legge di stabilità 2015 e dal nuovo regolamento di organizzazione dell'intero apparato ministeriale - di approntare le misure necessarie a individuare i soggetti funzionalmente competenti alla definizione del procedimento decisionale di spesa, a delinearne i compiti e a definirne i rapporti con l'amministrazione centrale. A ciò va aggiunto come, nella prospettiva di assicurare sul territorio la continuità dei servizi in precedenza svolti dal personale dei Comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, sia stata prevista la possibilità di continuare ad avvalersi del medesimo personale, sulla base di accordi o convenzioni. da ultimo, sottolineato come il Ministero della giustizia sia attivamente impegnato anche nella promozione delle attività formative dei soggetti coinvolti nel procedimento di spesa, coerentemente alle iniziative assunte dalla Scuola superiore della magistratura. Ed è proprio grazie al sostegno dei Comuni e alle sinergie sviluppate in sede locale che la transizione si è svolta senza evidenziare particolari disservizi, pur con le inevitabili difficoltà che il cambiamento ha comportato. Nel passaggio al nuovo modello di gestione si iscrive, pertanto, la definizione dei contributi ancora dovuti ai Comuni in virtù della pregressa gestione diretta della spesa. Preme, al riguardo, sottolineare che proprio la prospettiva di un corretto avvio del nuovo sistema delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari ha orientato l'impegno del Ministero nel regolare, definitivamente e al più presto, le posizioni pregresse con i Comuni, nel quadro legislativo di riferimento e con i limiti finanziari dettati dalle disposizioni normative che hanno regolato la quantificazione e la liquidazione dei rimborsi. Presidente della Repubblica n. 187 del 1998, difatti, la determinazione del contributo da erogare ai Comuni doveva essere assunta, annualmente, con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute. Con il fine di allineare le scelte di politica economico-finanziaria ai generali obiettivi di contenimento della spesa pubblica fissati anche in ambito comunitario, il decreto-legge n. 95 del 6 aveva previsto per il Ministero della giustizia risparmi in misura non inferiore a 30 milioni di euro per l'anno 2012 e a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, in termini di minori contributi ai Comuni per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Nel delineato quadro normativo, i tempi e l'entità dei contributi erogabili sono stati essenzialmente condizionati dalle misure di risparmio previste dal citato decreto-legge: oltre a doversi attendere che le spese fossero indicate a consuntivo dei bilanci comunali e sottoposte al vaglio delle commissioni di manutenzione, la liquidazione doveva essere successivamente disposta con decreto interministeriale e secondo rigide percentuali di rimborso. Con riferimento ai crediti maturati dai Comuni per l'anno 2012, dalle informazioni assunte presso il Ministero dell'economia e delle finanze e attraverso le competenti articolazioni ministeriali, consta come il decreto interministeriale abbia reso disponibile una somma pari a circa 77 milioni di euro, da imputarsi all'esercizio finanziario 2013. Per lo stesso esercizio era già stato erogato, con decreto del competente direttore generale di questo Dicastero del 5 marzo 2014, un acconto pari a circa 65 milioni di euro. Lo stesso decreto interministeriale ha determinato, in circa il 25,88 per cento delle spese effettivamente sostenute dai Comuni, la misura del rimborso liquidabile. Con decreto del direttore generale di questo Dicastero del 7 dicembre 2015 si è pertanto provveduto all'erogazione del saldo e, per alcuni Comuni, è stata operata la decurtazione degli importi risultati degli importi risultati eccedenti rispetto al contributo effettivamente determinato, erogati in acconto per le annualità precedenti. Anche il decreto per le spese sostenute nell'anno 2013 è stato firmato dai tre Ministri competenti ed è stato pertanto liquidato il relativo saldo. Per venire incontro alle difficoltà rappresentate dai Comuni, la direzione generale delle risorse ha disposto, con decreto assunto in data 12 febbraio 2016, l'erogazione dell'acconto per le spese sostenute nell'anno 2014, determinato secondo i parametri relativi al contributo liquidato, in via definitiva, per l'anno 2012. Il decreto interministeriale di determinazione del contributo spettante ai Comuni per l'anno di spesa 2014 è già stato sottoposto alla firma del Ministro della giustizia ed è attualmente alla firma del Ministro dell'interno e successivamente sarà trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze. Non appena completato quest'ultimo adempimento, si procederà alla erogazione ai Comuni aventi diritto del saldo spettante. Al fine della determinazione dei contributi spettanti fino al 31 agosto 2015, si sta invece procedendo all'esame dei rendiconti dei Comuni. Lo stanziamento di bilancio nello stato di previsione del Ministero della giustizia è pari, inoltre, a 111 milioni di euro per il 2014 e a 133 milioni di euro per il 2015. Dal 1° settembre 2015, alla luce di quanto disposto dalla legge di stabilità per il 2015, per il pagamento dei canoni, così come per le altre spese degli uffici giudiziari, sono state delegate le Corti d'appello. Nel quadro così delineato, i contributi erogati al Comune di Bologna per le spese sostenute per gli uffici giudiziari, sono i seguenti: per l'anno 2012 il Comune di Bologna ha ricevuto un contributo pari a 2.836.045,87 euro, euro, ripartito in 2.720.232,14 euro di acconto e 115.813,73 euro per saldo, a fronte di un rendiconto, al netto dei rilievi, pari a 10.958.446,18 euro. Per la determinazione del contributo è stata applicata la percentuale del 25,88 per cento che, come già evidenziato, è stabilita a livello nazionale tenendo conto, oltre che delle somme relative ai rendiconti trasmessi, anche dello stanziamento sul capitolo per l'anno finanziario di riferimento. Per l'anno 2013, il Comune di Bologna ha ricevuto un contributo pari a euro 3.613.507,38,

pari a euro 10.050.779,15. Per la determinazione del contributo è stata applicata la percentuale del 35,952 Per l'anno 2014, a fronte di un rendiconto presentato dal Comune di Bologna, al netto dei rilievi, pari a euro 9.423.746,72, è stato determinato il contributo nella misura di euro

Per l'anno 2015, fino alla data del 31 agosto 2015, anche il contributo dovuto al Comune di Bologna non è ancora determinato né determinabile, in attesa dell'esame complessivo dei rendiconti. Alla luce dei dati esposti, si intende rassicurare che saranno poste in essere tutte le iniziative che possano soddisfare, nella misura più adeguata, le aspettative dei Comuni sede degli uffici giudiziari. Nell'ambito dei lavori preparatori della manovra di finanza pubblica per il 2017-2019, sono, infine, all'esame del Governo iniziative finalizzate ad assicurare risorse, per l'importo complessivo di circa 300 milioni di euro, destinate al ripianamento del debito complessivo residuo verso i Comuni per il rimborso delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari sino al 31 agosto 2015.

un dato molto importante che sana una situazione veramente molto atipica, perché si imputavano ai Comuni spese che di fatto non erano di loro competenza.

la partita dei rimborsi ai Comuni per spese precedentemente anticipate. Vorrei infatti ricordare che, se la legge n. 190 del 2014, cioè quella che riporta in capo al Ministero della giustizia il sostenimento delle spese per gli uffici giudiziari, è entrata in vigore il 1° settembre 2015, rimangono ancora dei debiti pregressi da saldare confronti dei Comuni.

La legge del 1941 chiedeva ai Comuni non di sostenere, ma di anticipare delle spese che erano di competenza del Governo. L'articolo 110 della Costituzione parla chiaro quando dice che il funzionamento degli uffici giudiziari è di competenza Fino a qualche anno fa, queste spese venivano rimborsate in una misura che oscillava intorno all'80 per cento, e quindi mai integralmente, ma in una misura adeguata a coprire sostanzialmente la spesa anticipata, chiedendo comunque ai Comuni sedi di uffici giudiziari uno sforzo per la copertura piena di quella cifra, che spesso poi in realtà si riduceva magari ad affitti nominativi non saldati. Ma, a seguito di provvedimenti il cui avvio non è imputabile certo a questo Governo (la legge n. 95 del 2012, che prima il sottosegretario Migliore citava, è la legge sulla *spending review* firmata dal Governo Monti) e, nel momento in cui il Paese ha deciso di mettere mano ai conti pubblici e di attivare misure stringenti di revisione della spesa, si è attivato un meccanismo che io continuo a trovare improprio. Si sono, cioè, tagliati i fondi al Ministero della giustizia perché potesse coprire gli anticipi dei Comuni, portando il rimborso di quelle spese alle misure che il sottosegretario Migliore citava prima: nel 2013, 44 per cento nel 2014. Il resto di dette cifre è rimasta una spesa non coperta da parte dei Comuni. scaturisce anche la differenza fra un debito che, rispetto alle casse dei Comuni, è quantificato in cifre sostanziose (il comune di Bologna parla di 40 milioni dovuti dal Ministero della giustizia) e una quantificazione molto ridotta

Il Comune di Bologna - è stato il motivo che mi ha spinto a presentare questa nuova interrogazione su un tema su cui avevo già interrogato più volte il Governo precedentemente

è stata sanata dal punto di vista normativo una situazione impropria, che determinava uno slittamento di competenze fra lo Stato e gli enti locali, e così come, rispetto alla sostanziosa cifra

determinazione con cui il Ministero della giustizia in questi anni ha provveduto a efficientare la macchina della giustizia, sia dal punto di vista sia organizzativo e amministrativo, sia della revisione normativa

Credo che un contenzioso al TAR fra un Comune e il Governo sia una modalità irrituale che la politica dovrebbe riuscire